Comunico che è stato deferito ieri, in sede deliberante, alla 1a Commissione permanente il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente l'uso del *computer* nelle prove scritte per l'esame di giornalista (1939). La Commissione giustizia ha già espresso il proprio parere. La Commissione affari costituzionali è autorizzata a convocarsi in sede deliberante per l'esame del predetto provvedimento domani mattina, a conclusione del voto di fiducia, subito dopo lo svolgimento delle votazioni elettroniche previste sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sulle proposte della Giunta in tema di reati ministeriali. Inoltre, in relazione ad altre richieste pervenute alla Presidenza da parte di Presidenti di Commissione, sono autorizzate a convocarsi, nell'orario predetto, le Commissioni permanenti che lo ritengano necessario per l'esame di questioni di particolare urgenza.

signori del Governo, so bene che anche questa volta gli italiani dovranno rassegnarsi: questa indigestione di voti di fiducia, quattro in poche ore, non lascerà certamente spazio né ai dissidenti, né tantomeno alla protesta. "Abbaiano alla luna"; sorriderete voi del Governo a proposito di un'opposizione che ormai cerca disperatamente di evidenziare quanto siate evidentemente responsabili del disastro e della devastazione del Paese. Allora, signori del Governo, consentite brevemente anche a me di abbaiare alla luna. Nemmeno ascolterete, ma sentirà chiaro e forte la gente, la maggioranza degli italiani che non ne può più, che festeggerebbe la fine di questo Esecutivo con i *boatos* di piazza e che giustamente vi imputa la responsabilità di una terribile recessione, di una crescita da livello zero, di un'assenza di prospettive che mai aveva interessato così pesantemente il Paese. Li avete scontentati tutti: categorie, famiglie, singoli cittadini; mai un Governo aveva ravuto un'opinione pubblica così ostile e anche le categorie che da Presidente della Commissione difesa rappresento idealmente, quelle degli uomini in divisa, non hanno di che rallegrarsi. In Commissione difesa abbiamo rimandato due volte indietro la finanziaria con voto contrario ad un provvedimento che non individua risorse per uomini ai quali il Paese chiede la rappresentanza internazionale nelle missioni di pace, la sicurezza contro la criminalità organizzata, la sicurezza dei confini; uomini ai quali chiedete molto, ma ai quali sistematicamente date pochissimo. Sapere che questo Governo ha lasciato gli uomini in divisa senza nemmeno l'indispensabile, mi

*(Misto-SC)*. Signor Presidente, a differenza del collega che mi ha preceduto, do la mia totale disapprovazione politica e morale ad una finanziaria che riserva più di 23 miliardi per le spese militari e per massicci acquisti di armi offensive da guerra. La scelta di impegnare sempre più il Paese in un ruolo di grande potenza, che fa valere i suoi interessi in giro per il mondo, come ribadito peraltro purtroppo anche dal Capo dello Stato quando ha affermato l'intangibilità della costruzione della base di Vicenza e la lunga permanenza dell'Italia nella guerra in Afghanistan, credo cozzi contro i princìpi costituzionali. Inoltre, vi è la mia totale opposizione sul mantenimento ed allargamento di ingenti privilegi e detassazioni per imprese e banche, a scapito del risarcimento sociale e voltando le spalle alle attese ed ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

così palesemente trascurava gli aspetti più elementari della sicurezza - hanno ricevuto nel 2007 ben 20 milioni di euro tramite il cuneo fiscale. E così sarà anche per i prossimi anni, non avendo modificato, come da me proposto, la norma della vecchia finanziaria. Ovviamente il mio "no" alla fiducia richiesta è del tutto opposto a quello delle destre. È da un punto di vista di opposizione di sinistra, come peraltro la natura degli emendamenti che avevo proposto

Il voto del Movimento politico dei cittadini sulla finanziaria sarebbe di astensione perché non condividiamo alcuni aspetti già erano nei nostri deliberati del Senato ed altri che sono stati infilati sotto il tappeto alla Camera: alcuni veramente indigesti di fronte alle condizioni economiche con cui molti cittadini stanno affrontando queste festività. Tra l'altro, contrariamente a dichiarazioni del ministro D'Alema sulla finanziaria dell'anno precedente, secondo cui i lavoratori avrebbero visto in busta paga gli aumenti, i lavoratori ci han guardato e ci sono delle riduzioni: proprio una presa totale per i fondelli!

finanziamenti che dovrebbero andare ai pendolari vanno alla TAV; si finanzia la metropolitana perché i nomi sono belli ed altisonanti. Se qualcuno della Commissione trasporti va a Firenze a vedere il nuovo muro di Berlino che viene costruito, più basso ovviamente,

di riduzione della spesa e poi per un progetto si assume personale, addirittura c'è un passaggio dove si parla di 15 persone, di cui 3 o 4 dirigenti: non cavano i nomi,

senatori, ci apprestiamo a dare il nostro voto favorevole alla legge finanziaria per il 2008, così come daremo un voto favorevole sul disegno di legge in materia previdenziale. Con questo però consideriamo conclusa una fase della vita politica nazionale. Una fase che ha avuto alcuni meriti: è stata interrotta l'ormai settennale tendenza alla crescita della spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo; si interromperà la tendenza alla crescita della pressione fiscale. I conti 2007 chiuderanno probabilmente meglio rispetto a quanto atteso. Non è poco, ma non basta. Non basta per arrestare la tendenza al declino economico e civile. Non basta per ricostruire nel Paese la fiducia in se stesso e nelle sue istituzioni. Ancora in questa finanziaria vi è traccia di un atteggiamento che vede nella spesa pubblica uno strumento per la risoluzione dei problemi; dimenticando che in Italia la spesa pubblica è una parte rilevante del problema. Ancora una volta i benefici derivanti dalla crescita delle entrate pubbliche vengono dispersi in mille rivoli, senza avviare quella generalizzata riduzione delle tasse essenziale per rilanciare lo sviluppo e migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini. Molti servizi pubblici - sanità, trasporti, sicurezza - continuano a deteriorarsi. La pubblica amministrazione viene lasciata affogare nell'inefficienza e nello spreco. Neanche al culmine di una fase congiunturale espansiva il nostro bilancio pubblico raggiunge l'agognato pareggio; continua ad essere alimentato quel debito pubblico che costituisce la fornace nella quale il Paese brucia le proprie speranze in un futuro migliore. La questione non è semplicemente quella di accelerare una marcia fin qui troppo lenta e impacciata. In molti casi si tratta di cambiare la direzione verso la quale ci muoviamo. Noi non intendiamo mettere la testa sotto la sabbia per non vedere il declino dell'Italia; non vogliamo nasconderci la perdita di posizioni in ogni graduatoria internazionale; non ci rassegniamo a una condizione economica che vede la produttività del nostro lavoro stagnante, e con essa il salario dei nostri lavoratori. Siamo convinti che una serie coordinata di politiche - economiche, sociali, istituzionali - possa invertire le tendenze presenti. Siamo convinti che queste politiche debbano essere ispirate ai princìpi liberali: se ciascuno sarà più libero di perseguire il proprio disegno di vita - civile, economica, sociale - allora molto verrà da sé. Ma questa libertà non sarà possibile senza una decisa azione politica che riduca la spesa pubblica, riduca le tasse, riduca l'eccessiva ingerenza dello Stato nei molti campi dell'agire umano.

il Senato si appresta a licenziare la legge finanziaria 2008, un atto di Governo fondamentale nel suo esame combinato con i relativi provvedimenti collegati. Un atto coerente con il programma presentato agli elettori; un atto, soprattutto, fondamentale e necessario per il processo di ripresa dell'economia italiana. Tutto questo nell'ottica di una più equa distribuzione della ricchezza ai cittadini. Prima di entrare nel merito delle misure più rilevanti del provvedimento, vorrei brevemente fare accenno all*'iter* di questa legge, certamente tortuoso ma che non pare connotato, come l'opposizione vuol far credere, da tratti negativi. È, anzitutto, doveroso apprezzare il fatto che, dopo tanti anni, le Commissioni bilancio di Senato e Camera abbiano concluso i propri lavori con serietà ed approfondimento. Non sono, infatti, mancati i momenti di dibattito e di serrato confronto, anche durante la prima lettura del provvedimento in questa Assemblea, i cui numeri sono ben noti. Nonostante ciò, si è discusso articolo per articolo, emendamento per emendamento e il Senato ha saputo licenziare il provvedimento senza alcuna blindatura. Appare, pertanto, strumentale la critica mossa dal centro-destra circa il mancato rispetto delle prerogative del Parlamento, specie se si rievoca la prassi invalsa nella passata legislatura, in base alla quale il Governo bloccava ogni testo di finanziaria, nonostante i numeri che sorreggevano l'allora maggioranza in entrambe le Assemblee. La fase democratica di discussione è stata, in questo caso, ampiamente rispettata e oggi il ricorso alla fiducia è necessario soltanto per una questione di tempi. Certamente non si può fare a meno di notare come nel primo passaggio al Senato e successivamente alla Camera sia via via cresciuto il numero dei commi e degli articoli dello snello disegno di legge finanziaria presentato dal Governo. Il contenuto della legge si è dilatato con la produzione inevitabile di effetti distorsivi rispetto alla coerenza del provvedimento e alla chiarezza del testo. Tutto ciò mostra ancora una volta con evidenza la necessità impellente di intervenire sulla disciplina che definisce il contenuto dei provvedimenti presentati nell'ambito della sessione di bilancio, nonché sui meccanismi procedurali che ne regolano l'esame. Proprio in tal senso si muove il disegno di legge presentato dal Gruppo dei Popolari-Udeur, che dunque appare meritevole di sollecita calendarizzazione.

contenute nella legge finanziaria 2008. Concludendo, il Gruppo dei Popolari-Udeur esprime convinto il proprio voto favorevole alla fiducia posta dal Governo sui tre articoli che compongono il provvedimento.

ha prodotto oggi uno studio dal quale risulta che il 51 per cento degli italiani quest'anno non ha potuto risparmiare un centesimo. È il punto più basso mai toccato dal popolo italiano: un popolo che si è distinto e contraddistinto negli anni per essere il più risparmiatore del mondo. Spesso gli italiani sono passati all'estero per cicale, quando per lunghi decenni sono stati i sacrifici degli italiani che, con i loro risparmi, hanno fatto crescere benessere e produttività e fatto diventare l'Italia il grande Paese partecipe partecipe del G8. Oggi il nostro è un popolo distrutto, affamato; il popolo italiano, che poteva sicuramente sperare in un Governo dove la presenza delle tradizionali forze di sinistra avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento per la tutela dei più deboli e delle classi meno abbienti, si è ritrovato, invece, da questo Governo che ha addirittura due partiti comunisti al proprio interno, ad essere affamato, ad essere più povero, ad avere addirittura difficoltà a comperare un chilo di pane, visto che ormai arrivare al 20 del mese è un'impresa sempre più difficile. Dunque, siamo il ventre molle dell'Europa, l'Italia è il Paese più povero e più insicuro d'Europa. Noi speriamo veramente che, di fiducia in fiducia, si sia arrivati alle ultime fasi che questo Governo levi le tende, perché non siamo di fronte ad un problema di sopravvivenza ma ad un problema etico, morale. Noi speriamo che si vada presto al voto per consentire

Signor Presidente, siamo chiamati oggi ad esprimere il nostro voto sulla fiducia posta dal Governo per l'approvazione della manovra finanziaria. Il voto dell'Unione Democratica, che esprimo anche per il collega Bordon, sarà oggi un voto poliedrico, ricco di sfaccettature. Vi è, infatti, un'adesione convinta ed entusiastica per quella parte di manovra che ci ha visto promotori di una grande innovazione: il testo finale della norma sulla *class action*, concordato punto per punto con il Governo nell'evoluzione alla Camera (di ciò rendo merito al sottosegretario D'Andrea), è il massimo risultato che si poteva raggiungere nelle condizioni date. Con essa si rende effettiva la tutela dei consumatori e degli utenti, recependo nell'ordinamento italiano uno strumento che consente di collegare ad un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande o pretese individuali originate da un unico fatto illecito, estendendo gli effetti della decisione a tutti i soggetti che l'hanno chiesto. Vi è poi, signor Ministro, un'adesione perplessa e problematica per le condizioni generali di un Paese che soffre di troppe patologie (dalle morti bianche alla mancanza di prospettiva di sviluppo, dalla scarsa competitività alla debolezza salariale) per le quali questa manovra finanziaria non riesce a proporre interventi efficaci. C'è, infine, un'adesione responsabile, ma tormentata, per lo strumento utilizzato, la triplice fiducia, che testimonia la debolezza congenita di un Governo che non può tirare a campare senza una maggioranza politica. Con il voto di oggi si chiude per noi il periodo dell'irresponsabilità. Da gennaio, ogni forza politica dovrà dichiarare le sue reali intenzioni. Anche noi saremo pronti a farlo,

il Gruppo Socialista, piccolo ma significativo al Senato, annuncia il voto favorevole, ma per una questione di lealtà politica, perché la nostra cultura ed educazione civica

sarebbero molto ampie e potrebbero spingerci anche a un voto diverso. Oggi prevale la lealtà politica: dal prossimo anno prevarrà il merito. In questo provvedimento, come negli altri a questo collegato (il decreto sull'extragettito

l'indennità di inserimento al lavoro subordinata a piani di formazione per i lavoratori precari; ma ciò non è sufficiente, poiché continuiamo nella linea delle politiche occasionali. I Socialisti non sono d'accordo. Sul piano delle politiche fiscali, vogliamo e chiediamo politiche strutturali premiali, che si orientino a incentivare le imprese che investono in competitività. Compatibilmente con l'equilibrio di conti pubblici, avremmo preferito che l'extragettito fosse destinato all'abbattimento del debito pubblico. Vorremmo politiche di *welfare* universali, come negli altri Paesi europei. Vorremmo inoltre che ci si occupasse dei salari e del potere d'acquisto dei lavoratori una maggioranza di Governo e un Partito Democratico che lo fa molto con le chiacchiere e poco con i fatti. Perché, mi chiedo, signor Presidente, non tassare l'intermediazione in questo Paese?

C'è assenza di politiche strutturali e di capacità della politica di decidere. Ci sarà, e finisco, Presidente, poiché il tempo da lei assegnato non mi consente di andare oltre, un motivo per cui la Spagna, ancora prima di quanto Zapatero prevedesse, ci ha superato nel PIL pro capite.

è una fiducia a termine. Adesso basta. Abbiamo poche risorse; utilizziamole per politiche strutturali, non più per occasionali erogazioni, reversibili l'anno successivo per poi darle a qualche altra categoria. I Socialisti non seguiranno più questa linea. La lealtà politica questa volta prevale, ma dalla prossima volta prevarrà il merito per l'equità e la giustizia sociale di questo Paese. *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi del Governo, onorevoli colleghi senatori, in questa XV legislatura ho votato a più riprese la fiducia al Governo presieduto dall'onorevole Romano Prodi. L'ho fatto talora per convinzione, talora per senso di responsabilità, anche allo scopo di consentire all'Esecutivo un arco di tempo capace di permettere e garantire un efficace dispiegarsi dell'azione di Governo. Oggi, tuttavia, debbo registrare che una vastissima successione di insipienze, scelte improvvide ed errori tecnici giuridici costella il percorso della vita dell'Esecutivo. Di più: si moltiplicano le modalità tattiche tese a rassicurare di volta in volta i diversi segmenti della maggioranza parlamentare mediante un uso singolare e spregiudicato della produzione legislativa, talché si concede qualcosa ad un versante in un testo normativo e qualcos'altro, a mo' di compensazione, ad un altro versante dello schieramento di maggioranza in un altro testo normativo, con il risultato che a più riprese si sono dovute constatare contraddizioni e ambiguità in molti provvedimenti di legge. Tutto ciò mi induce, per senso di responsabilità verso la Nazione, alla decisione che mi appresto ad annunciare. So perfettamente che le condizioni in cui versa il centro‑destra non gli consentono di rappresentare oggi un'alternativa ministeriale seria e credibile. D'altro canto, non è affatto detto che un'eventuale crisi di Governo abbia come automatica conseguenza lo scioglimento delle Camere. Il Capo dello Stato ha a sua disposizione una molteplicità di scelte, non escluso il conferimento al presidente Prodi dell'incarico di formare un nuovo Governo o anche altre soluzioni che, nella sua saggezza istituzionale, il presidente Napolitano vorrà autonomamente valutare. Da ultimo, mi si consenta di sottolineare che, per un verso, l'aggravio e gli squilibri distributivi della finanza pubblica, per un altro verso gli ostacoli variamente frapposti sulla strada di un ragionevole dialogo tra le due principali forze politiche del Paese - e ciò dico indipendentemente dalla ipotetica scelta di questa o quella formula elettorale sono ulteriori elementi che confortano la mia sofferta decisione politica, che è la seguente: voterò oggi e domani la fiducia come puro e semplice espediente tecnico per evitare l'esercizio provvisorio, ma sia chiaro che il rapporto di fiducia politica con il Governo in carica si è per me esaurito, senza possibilità di recupero. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il voto di fiducia che ci apprestiamo a dare è particolarmente importante in quanto con esso prospettiamo e delineiamo al Paese quello che sarà il suo futuro prossimo. Questo voto rappresenta, infatti, il punto più alto di un percorso politico-legislativo di un anno e, al tempo stesso, quel percorso di orientamento delle finanze verso la crescita, il risanamento e l'equità, cioè verso i cardini principali del programma politico sul quale l'attuale maggioranza ha ricevuto il voto maggioritario dei cittadini.

proprio quelle correnti calde che stanno attraversando oggi la nostra società. La manovra che questo ramo del Parlamento si appresta ad approvare e sulla quale il Governo ha posto la fiducia prevede, tra l'altro, che le risorse finanziarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale vengano utilizzate per gli sgravi sulla casa e in favore delle fasce non autosufficienti e di quelle deboli. Più in generale, essa non fa altro che interpretare fino in fondo le esigenze del nostro Paese. Penso al fondo in favore delle persone non autosufficienti, allo stanziamento del piano straordinario per i servizi per i servizi socio-educativi e per il sistema integrato, per gli asili nido, nonché al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e al sostegno ai cittadini a basso reddito e a ciascun componente del nucleo familiare. Tutto ciò è un aiuto economico che deriva in parte dalle risorse ottenute grazie al recupero dell'evasione fiscale. Il pilastro riformista che questa manovra finanziaria adotta, così interpretando davvero i sentimenti dei nostri cittadini, è quello di affrontare con decisione ed in maniera non propagandistica il problema del costo della politica tanto caro al partito dell'Italia dei Valori - intervenendo su due piani. Anzitutto, perché la scelta di riclassificazione del bilancio, pur riducendo il grado di dettaglio della decisione parlamentare, consente contemporaneamente maggiore trasparenza e completezza nelle scelte di spesa operate, indicando così ai nostri cittadini, degli anni scorsi, in che modo e nel perseguimento di quali fini i soldi di tutti verranno spesi. Il primo piano è, quindi, quello della trasparenza, che passa, in primo luogo, attraverso la riqualificazione della spesa pubblica e poi attraverso numerose norme di misura che, a regime, comporteranno risparmi di notevole entità. Penso, per esempio, alla riduzione del numero dei Ministri e dei Sottosegretari, al taglio dei rimborsi elettorali, alla riduzione degli incarichi e delle consulenze nella pubblica amministrazione, alla riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali e degli assessori comunali; per non parlare poi, come è a tutti noto, della sospensione per cinque anni dell'aumento automatico dell'indennità di noi parlamentari. Sono tutte misure molto attese dai cittadini. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la manovra che ci apprestiamo ad approvare per il triennio 2008-2011 apre una nuova fase del nostro Paese e si fa carico davvero in maniera non retorica delle aspettative dei nostri elettori. Non resta che continuare così,

capire, ministro Chiti, che il Governo cade oggi, ma ancora non sentiamo lo schianto. C'è tempo per il botto.

Se fossi un giornalista titolerei: «Il Governo è caduto, ma ancora non ha toccato terra». Siete in volo ma, conoscendo la pesantezza di questo Governo, non mancherà molto allo schianto.

rationem*. Chiedo al Presidente della Repubblica se ci sono spazi per trovare un momento di equilibrio e ridare un nuovo Governo a questo Paese, o attraverso quello strumento o attraverso altro strumento parlamentare,

Le nostre chiacchiere rischiano di essere soltanto ancora più irritanti per chi ci ascolta. Prendiamo atto di quanto hanno sostenuto qui una decina di senatori che rappresentano oggettivamente quella differenza abbondante

solo per trovare un equilibrio per il Paese vedo come seconda ipotesi le elezioni immediate. Certamente, dopo le parole dei colleghi, non possiamo nascondere ancora una volta, come gli struzzi, la testa sotto la sabbia. la necessità, altrimenti avrebbero ragione a parlare di casta, di prendere responsabilmente in mano il problema principale, che è il fatto che questo Governo non vuole, nel Paese prima di tutto, e poi nel Senato e nella maggioranza, prenderne atto. Auguriamoci per le feste natalizie, anzi per il Santo Natale, tutto il bene possibile, ma facciamolo anche verso i cittadini italiani, dimostrando la grande responsabilità che abbiamo e concedendo al Presidente della Repubblica la la vostra visita prenatalizia allo stesso, di ridare al Paese un nuovo Governo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembrava proprio di sentire le campane funebri per questo Governo, ma mi sembra anche un po' troppo facile dire che noi avremmo chiesto, noi avremmo visto, noi avremmo preferito che la spesa pubblica fosse

perseguire con serietà l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Pagare 70 miliardi di euro all'anno solo di interessi è troppo per una comunità: è come se una famiglia, invece di comperare vestiti e libri di scuola per i bambini, dovesse portare tutto lo stipendio in banca. È troppo: questo deve rimanere, ma è anche giusto equilibrarlo rispondendo alle esigenze sociali che ci sono nel Paese. Pertanto, condividiamo l'impostazione di questa finanziaria, che ci sembra equilibrata e migliore delle altre. Siamo contenti che ci siano anche

sono state ulteriormente promosse le energie rinnovabili. È un segnale positivo. Penso, ad esempio, agli incentivi per la riqualificazione delle abitazioni, per i pannelli solari e per il risparmio energetico in generale. in generale. In questo contesto giudichiamo positivamente l'attenzione dedicata ai territori di confine, alle accise per il gasolio da riscaldamento e al teleriscaldamento con biomassa.

Sartori sul «Corriere della Sera» ha criticato il federalismo dicendo che si raddoppiano le spese. Certo che si raddoppiano le spese se la nuova Costituzione prevede che le competenze di una serie di settori debbano passare alle Regioni;

si prenda esempio. Se in certe zone del Paese si lavora bene, perché dovremmo schiacciarle e portarle verso il basso? Cerchiamo, siamo i primi promotori, se se possiamo, di mettere a disposizione le nostre esperienze, di promuovere tutto il Paese in questa direzione, dandogli un assetto molto più democratico, più vicino alla gente, con un federalismo vero che possa orientarsi ai bisogni della gente stessa e non

Paolo *(LNP)*. L'Aquila, 20 dicembre: la Guardia di finanza ha dovuto rinviare in Abruzzo operazioni di polizia giudiziaria urgenti perché mancavano soldi per la benzina delle auto. che ha rivelato il Comandante regionale delle Fiamme Gialle a margine della conferenza di bilancio. Il comandante ha precisato che si tratta di un fenomeno generalizzato in Italia, ma in Abruzzo si sono trovati spesso in difficoltà.

lotta all'evasione fiscale procede grazie al lavoro della Guardia di finanza che si lascia appiedata vuol dire fare affermazioni di maniera, superficiali ed inutili, peraltro, smentite quotidianamente. È un'agenzia di oggi, ma credo che in tutte le Province del nostro Paese dai rappresentanti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza

studiata, discussa, approvata al di fuori di questo ramo del Parlamento. Quindi, di quali riforme parli il Presidente del Consiglio in risposta alla giusta osservazione del presidente Napolitano non è dato sapere. Per quanto riguarda questa finanziaria, è evidente che una legge

sociale, economica e fiscale di un Governo e di una maggioranza che nella forma non riescono a dare le risposte che i cittadini si aspettano, meno che mai nella sostanza. Mi riferisco, ad esempio, all'ICI;

felici andrete a dire che, grazie al recupero dell'evasione fiscale, avrete trovato nuovi tesoretti da spendere e spandere in mille rivoli, lasciando comunque la Guardia di finanza sempre senza la benzina

ci troviamo di fronte a prospettive - ultimo elemento di analisi che consegue al DPEF - di crescita pessime, di aumento del debito pubblico. Lo sapete anche voi che le stime al ribasso del prodotto interno lordo sono impietose

Quindi, un PIL che crescerà in maniera molto contenuta, al di sotto degli altri Paesi europei, e un debito che continua a crescere. Ho sentito poco fa che state facendo la battaglia per la riduzione del debito pubblico; saranno scritti in qualche altra analisi, in qualche altro studio, ma in quelli che sono disponibili quotidianamente a livello europeo o nazionale non è così.

il 2008 vedrà costante il livello della pressione fiscale, anzi ritengo addirittura in aumento. Un Paese in declino;

questo Governo, questa maggioranza, ma anche i Governi e le maggioranze dei periodi passati hanno privilegiato sempre il concetto romanocentrico dell'economia e dell'attività legislativa, dimenticando quali sono le esigenze le necessità delle varie parti del Paese, quelle produttive, quelle che hanno sempre fino adesso mantenuto vivo il Paese sotto il profilo sociale, industriale, delle risorse previdenziali.

un Paese in declino che non riceve un minimo di risposte che tendano ad invertire questa pesante e pessima direzione che ha assunto; un Paese le cui componenti fondamentali - l'impresa, la famiglia, il territorio - sono svilite a fronte di interessi centralisti che consumano e drenano risorse, come è sempre stato fatto purtroppo in maniera diversa dai tempi dell'unità d'Italia, alla quale questo Governo, questa maggioranza,

in una situazione di grave crisi economica e sociale. Non parliamo poi della crisi dei valori alla quale il Paese è abbandonato, i valori della famiglia, i valori della sicurezza, quelli che ci dovrebbero far sentire comunità, che quotidianamente

Signor Presidente, onorevole sottosegretario Letta, onorevoli colleghi, il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, quando parla, credo che non sappia quello che dica oppure sa quel che dice ma non quel che fa;

Qui c'è già la prima bugia: con i cosiddetti "tesoretti" nell'anno 2007 sono stati finanziati 16 miliardi di maggiori spese, 7 miliardi e 400 milioni con il decreto-legge n. 81 e 8 miliardi e mezzo con il decreto-legge n. 159. Secondo esempio: si è affermato che ogni euro di maggiore entrata strutturale dovrà essere destinato alla riduzione della pressione fiscale. Qui la seconda bugia: la pressione fiscale è al 43 per cento, la più alta dal 1997, quando si entrò nel «club di Eurolandia», e tale resterà anche per il 2008. Terzo esempio. Si è affermato: ogni euro di maggiore entrata a carattere temporaneo dovrà essere destinato al miglioramento dei saldi di bilancio; riduzione del disavanzo e del debito pubblico. Ancora una volta terza bugia: le maggiori entrate, sia strutturali che temporanee, sono servite per finanziare una maggiore spesa pubblica che nel 2007 è cresciuta del 5,2 per cento rispetto al 2006, mentre il disavanzo è aumentato dall'1,8 per cento del PIL a legislazione vigente per arrivare al 2,5 È stato fatto l'esatto opposto di quello che era stato detto agli italiani. Il *deficit* pubblico è, quindi, aumentato: solo al Senato la maggioranza di centro-sinistra, per far quadrare i conti interni alla maggioranza e non certo quelli dello Stato, ha aumentato la spesa della finanziaria di altri 2 miliardi e 300 milioni rispetto agli 11 previsti. La spesa reale sarà molto più alta perché alcune misure non hanno una seria copertura finanziaria: parlo dei 20 milioni stanziati per sistemare definitivamente 200.000 precari della pubblica amministrazione a danno dei vincitori di concorso, dei giovani disoccupati e di quelli in attesa di mobilità. Parlo dell'eliminazione della quota esente dei *ticket* sanitari, che costa 860 milioni di euro a danno dei consumi intermedi, cioè della benzina per le volanti della polizia, degli affitti non pagati nelle caserme di Polizia e Carabinieri, delle fotocopiatrici senza *toner* dei tribunali e così via. Ma il danno si estende anche agli enti locali, soprattutto del Sud, che si vedono reinseriti nei vincoli del Patto di stabilità interno per gli investimenti fatti in cofinanziamento con i fondi europei. Parlo, infine, dell'assunzione dei dipendenti pubblici che saranno destinati al recupero dell'evasione fiscale per i quali è prevista la cosiddetta autocopertura finanziaria. Senatrici e senatori del centro-sinistra, nel 2008 avremo minori entrate permanenti che determineranno un maggior disavanzo, un aumento delle materie prime e del costo del petrolio che ha raggiunto la cifra *record* di 100 dollari al barile, un aumento dell'inflazione già al 2,3 per cento con riduzione del potere d'acquisto di stipendi e salari, una diminuzione dell'*export* a causa del cambio euro-dollaro che ha raggiunto la cifra *record* di 1,50, una diminuzione dei consumi interni a causa della riduzione del potere d'acquisto e della riduzione di disponibilità di reddito delle famiglie, un aumento della pressione fiscale per compensare le minori entrate che si registreranno a causa della stagnazione economica e, quindi, della minore crescita del PIL che è prevista crollare al di sotto dell'1,3 per cento; molti disinvestimenti verso l'area di influenza del dollaro con riduzione del tasso di competitività del nostro Paese, un aumento dei tassi di interesse della Banca centrale europea per fermare l'inflazione con relativo aumento del costo del danaro; un probabile aumento della tassazione dei capitali dal 12,50 al 20 per cento, con conseguente disinvestimento nelle società quotate, con dislocazione del risparmio risparmio dagli investimenti produttivi ad altre forme di speculazione finanziaria. Questo è lo scenario che gli italiani avranno di fronte nel 2008. Per esorcizzare tale scenario, il Governo ha due sole possibilità: una riduzione drastica della spesa pubblica in modo selettivo: salvaguardare cioè solo la spesa sociale, riguardante la scuola dell'obbligo, gli incentivi alla famiglia ed alla natalità; un punto centrale del programma di questo Governo sollecitato proprio dal sottosegretario Letta che per l'UDC, comunque, rimane una questione centrale. In secondo luogo, favorire e migliorare la produttività: la produttività per occupato in Italia, a parità di potere d'acquisto, è scesa molto più velocemente che nell'Europa a 27. La bassa produttività così come il tasso di disoccupazione e di occupazione sono strettamente legati alla rigidità del mercato del lavoro, le giovani età di prepensionamento e l'inefficienza del pubblico impiego. Per ridurre la spesa pubblica e migliorare la produttività occorre una grande capacità di concertazione tra Governo ed organizzazioni sindacali. Occorre uno scambio tra una efficace politica di salvaguardia dei redditi ed un nuovo patto per il lavoro e la produttività. C'è una parte del sindacato disponibile ma è interdetto da posizioni estremiste presenti nello stesso Governo. La verifica prevista a gennaio rafforzerà queste componenti chiederanno addirittura la cancellazione della legge Biagi. Come si può pensare di migliorare il sistema dei fattori totali, della produttività e competitività nazionale avendo ancora in testa la lotta di classe? Ha detto bene Dini, il 15 novembre scorso: questo Governo non appare adatto a realizzare le politiche necessarie per invertire la tendenza al declino economico e civile del nostro Paese. Un'altra sfida è l'utilizzo dell'attivo patrimoniale del nostro Paese, che rappresenta il 130 per cento del PIL. Si tratta di vendere parte della RAI, dell'Alitalia, dell'ENI, dell'ENEL, delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e della proprietà ANAS. Sono attività economiche di mercato, perché devono pesare sulla fiscalità generale? Perché la proprietà deve essere pubblica? Perché non devono competere con altri privati sul mercato dei servizi? Perché non deve valere anche per loro la regola qualità-prezzo, la regola della minima spesa e della massima resa? Se si potesse realizzare questo programma di modernizzazione si potrebbe ridurre della metà i 70 miliardi di euro che paghiamo ogni anno per gli interessi passivi sul debito pubblico. La globalizzazione, cari amici, ci costringe ad essere all'avanguardia in tutti i settori nei quali è forte l'intensificarsi della concorrenza. La globalizzazione porta con sé una modernizzazione permanente, che coinvolge imprese e politica. C'è da noi una sinistra che ama definirsi comunista, quando il comunismo nel mondo è scomparso in tutti i Paesi avanzati, perché hanno sconfitto la povertà con la libertà. Occorre in Italia una politica di modernizzazione. Bisogna pensare, decidere e fare. Occorre risolvere il problema della governabilità e di una politica che decida. Occorre cambiare le regole del gioco: legge elettorale senza rendite di posizione; riforme istituzionali; diversi poteri del *Premier*; diverso bicameralismo; nuovi Regolamenti parlamentari; semplificazione del quadro politico. Questa è la proposta dell'UDC. Occorre un Governo di responsabilità pubblica fondato su un patto istituzionale per le riforme strutturali, che governi per il tempo necessario all'approvazione delle riforme e vada poi al voto con nuove regole, che garantiscano l'alternanza bipolare, con coalizioni di programma. Le coalizioni, cari colleghi, sono forti quando sono omogenee, non quando sono numerose. Siamo consapevoli che il Governo Prodi non cadrà finché c'è la paura di nuove elezioni che riportino Berlusconi al Governo. Sappiamo anche però che un Governo diverso da quello attuale, che realizzi le riforme che servono al Paese, non è pensabile senza Berlusconi. Per uscire da questa condanna all'ingovernabilità è necessario che Prodi e Berlusconi favoriscano una soluzione diversa da loro per il bene dell'Italia: si dimetta Prodi; pensi all'Italia prima che a se stesso. Lo hanno detto, poco fa, i senatori Manzione e Fisichella: il Governo finisce sabato prossimo, con l'ultimo voto di fiducia sul *welfare*. Ormai la crisi è aperta. Per queste ragioni e con questa consapevolezza noi dell'UDC votiamo contro la fiducia a questo Governo, perché ogni giorno di più che vive il Governo Prodi è un giorno in meno per il bene dell'Italia. Noi dell'UDC stiamo lottando per costruire regole nuove, dove possa emergere un'Italia diversa, un'Italia migliore, un'Italia libera e democratica. *(Applausi

impegnati nella costruzione di una confederazione unitaria, voteranno la fiducia. Siamo convinti che, allo stato, non esista un'alternativa a questo Governo che non sia di peggioramento.

Poi, di fronte a scelte a volte non comprese, né condivise, c'è stata prima incredulità, poi è subentrata anche molta tensione. Ora avvertiamo preoccupati un appesantimento nei rapporti interni alla maggioranza e fra maggioranza e Governo e chiediamo proprio al Governo di operare con urgenza perché questo stato sia superato. Rispettiamo le aspirazioni del nostro elettorato, che non è di opinione; sono aspirazioni legittime e concrete: tiene al lavoro; non vuole che si muoia nelle fabbriche e nei cantieri; aspira ad un nuovo modello di sviluppo economico dettato dal rispetto della natura e dell'ambiente; accoglie, eguale fra gli uguali, ogni orientamento sessuale; aspira a liberare le donne da ogni subordinazione e violenza; vuole consegnare ai giovani una società laica, libera ed egualitaria. Il nostro giudizio di merito sulla finanziaria coglie aspetti importanti, positivi: la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione è la prima seria inversione di tendenza rispetto ad un mercato del lavoro massacrato dalla legge n. Ma questo segnale ha subito un colpo con il Protocollo sul *welfare* su cui, come il Governo sa, il nostro giudizio è fortemente critico e non rassegnato. Di fronte ad un'ondata micidiale contro i costi della politica (fatta di qualunquismo, certo, ma anche di rabbia popolare, che va ascoltata), abbiamo lavorato con successo perché nella finanziaria la riduzione non avvenisse a scapito della democrazia e non colpisse la rappresentanza popolare. È la prima volta, inoltre, che una finanziaria si misura seriamente con la questione ambientale, certo, forse in modo ancora insufficiente, ma infine l'ambiente non è trattato come un orpello, come un aggettivo da aggiungere all'inizio o alla fine di un periodo, ma come una grande questione, ché tale è. Allo sviluppo di questo Paese non servono opere faraoniche: serve un rapporto armonioso tra ricerca, innovazione tecnologica e di prodotto e rispetto per l'ambiente. Alla stragrande maggioranza delle persone interessa di più (mi creda il Governo) che funzionino i trasporti per i pendolari piuttosto che la TAV. Allo sviluppo del Paese non serve tagliare lo Stato sociale, ma, al contrario, renderlo sempre più accessibile a tutti e sempre più efficiente, cancellando le a volte mostruose differenze tra territori, tra Nord e Sud, tra centro e periferia. I nostri partiti, signori del Governo, hanno una cultura che li porta a valorizzare ogni passo in avanti. E qui li abbiamo valorizzati. Ma quella stessa cultura ci mostra in tutta la sua ampiezza l'insufficienza di una politica da cui l'elettorato si aspettava, e ancora si aspetta, cambiamenti radicali che accompagnino positivamente la vita delle persone dall'infanzia alla scuola, al lavoro, alla vecchiaia. Il Governo ha operato una forte azione di risanamento: bene, diciamo noi. Ha fatto una cosa mai accaduta nella storia della Repubblica (sfido chiunque a dire il contrario): ha combattuto e combatte, con ottimi risultati, l'elusione e l'evasione fiscale. che quando ero una giovane lavoratrice ed una giovane militante comunista le tesi congressuali del sindacato e del partito iniziavano sempre con parole sull'esigenza di combattere l'evasione fiscale come un fatto elementare di giustizia e di equità. Quelle parole le ho lette e le ho scritte in tanti di quei documenti che potrei ripeterle a memoria; quindi, non potremmo non apprezzare. Ma i lavoratori dipendenti e i pensionati ricevono ogni fine mese buste paga povere ed insufficienti da cui le tasse vengono tolte prima ancora che arrivino nelle loro tasche. Sono gli unici che senza evasione, senza elusione, le pagano tutte. È sulle loro tasse che si reggono, da sempre, il sistema sanitario, quello previdenziale, quello scolastico: voci di spesa, vengono chiamate. E da sempre, anche durante i lavori di quest'ultima finanziaria, c'è chi si mette di traverso, perché quelle spese frenerebbero lo sviluppo. Sono quelli che poi storcono la bocca di fronte alla lotta all'evasione e che civettano con le corporazioni. Noi condividiamo l'azione del Governo contro l'evasione e difendiamo il diritto di ognuno ad una pensione dignitosa, alla sanità ed alla scuola pubbliche, e con i soldi recuperati sarà necessario sgravare quelle buste paga povere ed insufficienti dei lavoratori e dei pensionati, con cui non si arriva alla fine del mese, dall'eccessivo peso delle tasse. Signori del Governo, noi avvertiamo una seria distanza fra il programma con cui l'Unione si è presentata alle elezioni e le vostre scelte politiche. Non si tratta solo di gradualità, che comprendiamo, accompagniamo. Si tratta della rotta che si prende, e spesso l'abbiamo considerata, ed è stata, sbagliata. C'è un buco nero in questa finanziaria. Le spese per gli armamenti sono fortemente aumentate. *(Applausi Che segnale è verso quella moltitudine di persone, laiche e cattoliche, dell'associazionismo e del volontariato, che manifestano e credono nella pace? Che senso ha continuare una guerra perduta come quella in Afghanistan o raddoppiare la base di Vicenza? Per quella base noi chiediamo una moratoria, signori del Governo. *(Applausi dai Gruppi* Noi vogliamo quell'Italia che ripudia la guerra, che non manda allo sbaraglio tanti giovani militari, che non si rende complice dell'uccisione di tanti civili innocenti, che non fa o che non rischia di fare del suo territorio una portaerei statunitense. La finanziaria distribuisce soldi ai redditi e alle classi più basse. Molto bene, diciamo noi, c'è tutto il nostro consenso; ma bisogna andare oltre.

in quest'Aula che pensa che un lavoratore precario possa avere quarant'anni di contributi o che pensa si possa campare con quei 400 euro, che, fra l'altro, non prenderà mai? Vedete, nella nostra maggioranza ci sono spesso polemiche, anche aspre, tra chi si adopererebbe per la famiglia e chi invece alla famiglia sarebbe ostile. La famiglia, luogo di mille contraddizioni e anche di dolori, persino di violenze, ha bisogno di essere aiutata, ha bisogno di servizi, di assistenza agli anziani e ai disabili. È sbagliato ed è anche crudele considerare famiglia solo quella che sceglie, perché vuole o può farlo, il matrimonio. La famiglia è il luogo degli affetti, dove le persone decidono di passare insieme la vita affrontando gioie e diversità. La famiglia non è un fatto ideologico: è qualcosa di profondamente e straordinariamente forte e concreto. Noi vi chiediamo, signori del Governo, che gli uomini e le donne che decidono di formare una famiglia, nel matrimonio o al di fuori di esso, sentano che questo Governo e la sua maggioranza gli sono amici. Ci aspettiamo politiche contro la discriminazione e a favore dello Stato di diritto.

signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, la francamente stiamo vivendo in quest'Aula una situazione surreale. Il Governo ha chiesto la fiducia e i Gruppi parlamentari dell'ex maggioranza dichiarano di votare per l'ultima volta la fiducia, motivando questo loro voto con critiche pesantissime, radicali allo stesso Governo e alle proposte contenute nello stesso provvedimento di legge finanziaria, sul quale il Governo ha chiesto la fiducia. Il problema è che questa situazione surreale è condita da un paradosso. Tale paradosso mi fa ricordare quel simpaticone, quel personaggio dei fumetti, meno noto di altri personaggi di fumetti: Orazio, il fidanzato di Clarabella. Francamente, in questo anno e mezzo, quasi due, di Governo, più volte il Ministro dell'economia, alla resa dei fatti, è apparso l'Orazio fidanzato di Clarabella. perché l'ultima che ha combinato il Ministro dell'economia pochi giorni fa è quella di aver annunciato che occorrerà per l'Italia

Forse, come spesso capitava ad Orazio, non si è reso conto che, nello stesso momento in cui faceva questo annuncio, presentava in Parlamento, a sua firma a firma dell'intero Governo, una manovra che complessivamente, da luglio fino a domani o a stasera, determina un aumento di 27,7 miliardi di spesa pubblica in più, lievitati a 31,3 miliardi dopo l'uscita del provvedimento dalla Camera e il rientro in quest'Aula del Senato. Il paradosso consiste quindi proprio nel chiedersi se il Ministro dell'economia, che guarda dal 2009 in poi, ha guardato i conti del 2007 e del 2008. Purtroppo, quella che stiamo vivendo in un clima surreale è palesemente una farsa, signor Presidente; una farsa per la quale il Governo otterrà un voto di fiducia su un testo per il quale ha chiesto la fiducia e che - molto pacatamente uno di quei banchetti dei *suk* delle città arabe dove c'è un pezzetto qua e un pezzetto là per tutti, un po' di più, un po' di meno. Altro che mercato, efficienza e concorrenza! La tecnica con la quale si ottiene questo voto di fiducia ultimativo è quella del *suk*. Non si negano 100.000 euro a nessuno, né 2 milioni di euro, né 3 milioni di euro:

al risanamento, il *deficit* pubblico (che nel 2006, al netto dei trucchi contabili e del falso in bilancio, era del 2,2 per cento del PIL) rischia di rimbalzare di nuovo verso il 3

per cento delle risorse viene palesemente assegnato alla maggioranza di riferimento di cui voi non fate parte e che sta fuori da quest'Aula (banche, grandi imprese, grandi interessi),

sono addirittura *una tantum*, come quello in favore degli incapienti. Ma dov'è la tragedia? La tragedia, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, la si legge nei numeri e rappresenta la grande occasione mancata per l'Italia in questo anno e mezzo di Governo Prodi. Cari colleghi, nel 2005 gli italiani pagarono 629 miliardi di tasse complessive come entrate della pubblica amministrazione; nel 2006, 663 miliardi; nel 2007, contrariamente a quanto falsamente detto dal Governo all'inizio dell'anno, 703 miliardi. Emersi i dati a fine anno, avranno pagato 730 miliardi di tasse e nelle previsioni 2008 pagheranno 770 miliardi di tasse, cioè

avremmo dovuto oggi portare a casa, maggioranza e opposizione, o ex maggioranza, forse ex opposizione, quanto meno o un'imponente e rapida riduzione del *deficit* e del debito pubblico, o un'imponente parziale riduzione della pressione fiscale, o entrambi. Invece, nello stesso periodo, la spesa pubblica complessiva, che era di 787 miliardi nel 2005, è balzata a 734 miliardi a 760 quest'anno e a 800-810 miliardi l'anno prossimo, con un disavanzo - come ho già detto - che rischierà di porci ancora sotto la lente di ingrandimento dell'Unione Europea, in un momento in cui la crescita economica rallenterà. Concludo, signor Presidente, con una osservazione. Più che motivare il voto contrario alla fiducia da parte di Alleanza Nazionale, ho voluto francamente sottolineare, cari colleghi, le tante ipocrisie con le quali i diversi Gruppi della ex maggioranza si riferiscono ad un Governo di minoranza, annunciando il loro voto di fiducia tecnica, e quindi la fine del Governo, su un altare preciso: meglio votare questa manovra che fa schifo a tutti, piuttosto che ricorrere all'esercizio provvisorio. Ebbene, la responsabilità politica e istituzionale vorrebbe che a questo punto - (e, purtroppo, lo debbo dire con sofferenza anche personale e professionale)

è necessaria, sia per questioni specificamente riguardanti la finanziaria, sia per il contesto istituzionale nel quale siamo oggi chiamati ad esprimere il nostro no di fiducia, stavolta - al Governo e non soltanto alla finanziaria. Per quel che riguarda le questioni economiche, già è stato detto bene e molto dai colleghi che mi hanno preceduto, ma sono necessarie forse alcune ulteriori precisazioni su questioni emerse proprio nel periodo in cui la legge finanziaria ha continuato il suo *iter* in Parlamento. Incredibilmente, il nodo della crescita che l'attuale Governo si era impegnato solennemente ad affrontare, non solo non è affrontato, ma - di fatto - già sancisce il fallimento della politica economica e finanziaria dell'Esecutivo. Mentre l'Italia già inesorabilmente ricomincia a crescere più lentamente, si nota che una tale progressiva erosione dei margini di crescita è in controtendenza,

la Spagna ci ha superati nel PIL *pro capite*, il che significa che la sua crescita in questi anni è stata di gran lunga superiore alla nostra e continua ad esserlo; nell'ambito degli altri Paesi dell'Unione Europea, l'Italia è ritornata ad essere il fanalino di coda. Dunque, la politica del Governo sul terreno della crescita ad oggi è fallita: non ci sono altre parole. Non renderemmo verità al Parlamento se non usassimo queste parole forti: la politica è fallita. Siamo di nuovo il fanalino di coda e lo siamo mentre gli altri crescono, senza parlare ovviamente dei Paesi più lontani da noi che crescono a ritmi addirittura strabilianti.

Alitalia è stata di un centesimo di euro per azione. È chiaro che in settori importanti come il trasporto aereo la valutazione della nostra compagnia si è ridotta

La cosa grave è che l'altra grande tendenza, relativa all'aumento delle entrate, si è ulteriormente consolidata in questo periodo. Siamo giunti ad un aumento delle entrate nel

le tredicesime della gente comune sono state ridotte; dunque, quando fate la retorica dei salari e degli stipendi bassi,

questo è francamente irritante, soprattutto se confrontato alla retorica che continuamente manifestate. Dicevo, non avete usato - lo ha detto bene prima di me il senatore Baldassarri - questo enorme aumento delle entrate né per una cospicua riduzione del debito, né per una cospicua riduzione della pressione fiscale, proprio per aggredire il nodo della crescita. Potevate farlo liberando risorse attraverso la riduzione del servizio del debito, potevate farlo attraverso una riduzione della pressione fiscale, potevate usare un *mix* tra due politiche di questo tipo: no! Avete invece usato tutto l'aumento delle entrate o gran parte di esso per un aumento della spesa corrente e, nel corso dell'*iter* della finanziaria, abbiamo visto che la spesa corrente che aumentate è quella strutturale e crescente nel tempo, il che significherà nuove rigidità nel bilancio, perché la spesa corrente è quella più rigida da ridurre. Ecco allora che fra qualche tempo potremmo trovarci di fronte ad una diminuzione delle entrate in conseguenza di una minore crescita e ad un aumento strutturale della spesa corrente che non riuscirete a finanziare se non con un ulteriore indebitamento e quindi con un peggioramento anche dei parametri di Maastricht. Veramente è tutto molto grave. Perché questo? Per una dissipazione clientelare che nell'ultima parte si è consolidata, questa sì, ed ha portato ad una finanziaria che era stata preannunciata come agile e snella, mentre direi che soffre della malattia del secolo dei Paesi ultramoderni, dei Paesi ultramoderni, cioè una obesità evidente: e, com'è noto, l'obesità normalmente nuoce, e tanto all'organismo, cioè alla Nazione. Infine, signor Presidente, il Capo dello Stato aveva lanciato un monito severo e assolutamente da accogliere: aveva detto di fare attenzione alle fiducie.

Lo testimonia il fatto che l'unico momento nel quale si è approvata una legge in Parlamento è stato al Senato, lì dove i numeri della maggioranza sono risicatissimi, se non inesistenti, e invece alla Camera, prima, e adesso di nuovo al Senato, la maggioranza deve porre la fiducia. Alla Camera, dove c'è una maggioranza enorme, il Governo ha dovuto mettere la fiducia e oggi la rinnova al Senato. Questo perché le contraddizioni interne percorrono e devastano la maggioranza e soltanto un atteggiamento serio dell'opposizione, come quello che c'è stato al Senato della Repubblica, ha consentito una normale dialettica parlamentare.

spero di no ma temo di sì, il Governo apporrà la fiducia. In questo caso il Senato della Repubblica, che ha mostrato sulla finanziaria di saper essere presidio della dialettica parlamentare, viene totalmente pretermesso. Noi non abbiamo avuto la possibilità di discutere, né in Commissione, né in Aula, una questione rilevantissima come il Protocollo sul *welfare*. Così si insidia seriamente, ripeto, seriamente ed ecco perché poi accadono quelle rincorse alla piccola spesa che hanno connotato questa finanziaria: perché non si consente al Parlamento di discutere e deliberare sui grandi temi dalla Nazione; ed il *welfare* è certamente uno di questi. troviamo di fronte ad una situazione istituzionale che ritengo ormai giunta ad un livello di gravità assoluta, per la quale, davvero, prima va via questo Governo e meglio è per tutti i cittadini italiani,

in cui si muovono sparute minoranze dinamiche sopraffatte da una montante marea di corporazioni che resistono all'innovazione e con ciò condannano l'intero organismo alla decadenza? Nascono dall'analisi di due caratteri della realtà socio-economica del Paese: l'inefficienza economica e la crescente disuguaglianza sociale, che si sono venute affermando come caratteri dominanti in questa ultima fase. Due caratteri che la storia economica di tutti i Paesi capitalistici avanzati conferma essere strettamente correlati tra di loro. Cipossono essere brevissimi periodi di grande sviluppo economico, cioè di grande crescita, in un contesto di crescente disuguaglianza sociale; ma presto o la tendenza alla disuguaglianza sociale si inverte, e allora la crescita si stabilizza, oppure il mantenimento di un elevato livello di disuguaglianza finisce per essere ostacolo insormontabile al mantenimento di un adeguato livello di crescita. È la storia dei Paesi industriali avanzati di questi due secoli. Da più dieci anni, per la precisione da tredici, colleghi dell'opposizione (e sarebbe bene che ci mettessimo d'accordo almeno su questi dati essenziali, non attribuendo il rischio di declino del Paese all'azione del Governo dei sei mesi precedenti, perché sarebbe un'offesa all'intelligenza di tutti, reciproca, nostra, vostra, chiunque lo faccia), reciproca, nostra, vostra, chiunque lo faccia), il prodotto per abitante cresce ad un ritmo inferiore a quello medio dell'Unione Europea e della stessa area dell'euro, che pure nel contesto delle macroaree che si confrontano nell'economia globale è quella cresciuta meno nel corso di quest'ultima fase. Ciò che è più importante, il prodotto per ora lavorata, negli ultimi tredici anni o non cresce affatto, come è accaduto nei primi anni 2000, o cresce meno di quanto accada nei Paesi dell'area dell'euro con cui noi ci confrontiamo, con il risultato che, ovviamente, anche quando cresce non èin grado di recuperare il *gap* che ha accumulato negli anni in cui non è cresciuto.

con l'aggravante, però, che mentre nel Regno Unito le politiche redistributive dei Governi laburisti di quest'ultimo decennio stanno intaccando il livello di povertà relativa, in Italia esso è assolutamente stabile e, colleghi, ciò che è più grave, per noi, ma credo anche per voi, assolutamente indifferente al susseguirsi dei Governi di centro-destra e di centro-sinistra. Siamo dunque un Paese poco dinamico e molto ingiusto, con lo Stato più indebitato dell'Occidente avanzato. Evidentemente, e da molti anni, l'elevato livello di spesa pubblica è assai poco correlato alle sue due canoniche giustificazioni fondamentali: come prima, quella per cui lo Stato spende per incentivare la crescita oltre i livelli raggiungibili senza quell'intervento dello Stato stesso;

In Italia, cari colleghi, spendiamo ogni anno di più come Stato, ma senza che questa spesa risulti capace di sostenere il ritmo dello sviluppo; ogni anno spendiamo di più ma senza che questa spesa aiuti chi sta più male a risollevarsi. Signor Presidente, quando noi formuliamo un giudizio positivo sulla legge finanziaria e di bilancio al nostro esame lo facciamo assumendo esplicitamente il punto di vista di chi sa che ogni azione di politica economica, ogni scelta di prelievo e di allocazione delle risorse, ogni iniziativa di riforma e ristrutturazione della macchina pubblica deve essere giudicata in rapporto alle seguenti elementari domande. domanda: serve per lo sviluppo questa misura che stiamo discutendo? Seconda: serve per una migliore redistribuzione del reddito e per aiutare chi sta peggio? Terza, se la risposta è affermativa ad entrambe le domande: il costo dell'intervento è sufficientemente basso così da non obbligare ad un *surplus* di prelievo fiscale?

noi senatori democratici rispondiamo che sì, emerge dal complesso di queste misure una linea di politica economica che nel difficilissimo contesto dato muove nella direzione di un recupero di capacità competitiva del sistema e consegue obiettivi di riequilibrio sociale senza pregiudicare la riacquisita stabilità della finanza pubblica. Riacquisita, colleghi dell'opposizione. Anche su questo le giaculatorie, le prediche le accettiamo, ma non da quel senatore Biondi).* In cinque anni, obiettivamente senatore Biondi, mi consenta - direbbe una personalità che le sta

Noi non siamo un granché, ma voi avete fatto un disastro. L'obiettivo della competitività ispira le scelte in materia di fiscalità d'impresa. A luglio 2007 tre punti in meno di cuneo fiscale e contributivo sul lavoro; nel 2008 cinque punti in meno di aliquota di prelievo sul reddito d'impresa e, per le imprese marginali, la più significativa delle azioni di semplificazione fiscale dai primi anni Una partita di giro - come ho sentito dire dai colleghi dell'opposizione - per le imprese tra minori aliquote ed allargamento della base imponibile. Niente di più infondato se ci si riferisce alla maggiore indeducibilità degli interessi passivi. Chiunque abbia mai visto un'impresa sa che basta cambiare i suoi comportamenti per approfittare della riduzione di aliquota e non pagare la penalizzazione dell'allargamento della base imponibile. Quanto agli ammortamenti anticipati, le correzioni adottate da Senato e Camera rendono la norma ampiamente sopportabile anche dalle imprese più innovative, mentre la norma sul trattamento fiscale della quota di salario da contrattazione decentrata apre uno spiraglio per una riforma del modello contrattuale che affronti finalmente la questione salariale anche dal lato della redistribuzione a favore dei lavoratori, dei vantaggi derivanti da incrementi di produttività. Anche in tema di politiche sociali si sono poste le premesse per una svolta rispetto ad una lunga fase nella quale prima i governi di centro-sinistra, poi i governi di centro‑destra hanno pensato di aiutare i più deboli agendo sul tasto delle detrazioni e deduzioni fiscali. Finalmente, sia pure con un accenno, le politiche fiscali contenute in questa manovra finanziaria assumono a riferimento prioritario gli incapienti, cioè quelli che non possono essere aiutati con detrazioni e deduzioni semplicemente perché di tasse non ne pagano perché troppo poveri. Ma per tornare alla domanda da cui sono partito e terminare: i costi della finanza pubblica, di questi interventi, sono tenuti sufficientemente bassi? Sul piano meramente contabile la risposta è si. Il relatore di maggioranza ha già dimostrato come siano infondate le tesi che qui pure sono state ripetute a proposito dell'esplosione della spesa pubblica che è in aumento, ma è compensata da una corrispondente riduzione di spesa. Questa è la legge finanziaria che abbiamo al nostro esame. però il nostro ragionamento deve andare dal presente al futuro di cui questa legge finanziaria delinea i contorni. Lo fa l'articolo 1, comma 4, laddove si dice che tutto l'eventuale extragettito - tutto e non solo quello derivante dalla lotta all'evasione fiscale dovrà essere impiegato per ridurre la pressione fiscale sui contribuenti leali. È una decisione di enorme rilievo che determina, per il Governo e il Parlamento, un vincolo di straordinaria portata: realizzare tutto l'aggiustamento dei conti necessario e finanziare qualsiasi nuova spesa con corrispondente riduzione di spesa. È possibile? I fallimenti del passato consigliano di non rispondere sì con faciloneria, a cuor leggero, a questa domanda. Ma qui si misurerà l'efficacia dei progetti di ristrutturazione delle forze politiche che sono in corso, sia nel centro‑sinistra che nel centro-destra, perché questo è un compito gravoso per il Paese di fronte al Paese. La politica non è stata in grado, in questi anni, di riqualificare e ridurre la spesa pubblica, perché è troppo debole in rapporto agli interessi che sono incistati nella spesa pubblica e resistono al cambiamento.

dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza. Ricordo che ciascun senatore, chiamato dal senatore segretario, dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato,

Castelli,

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza. Ricordo che ciascun senatore, chiamato dal senatore segretario, dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Micheloni, Molinari,

Villecco Calipari, Villone, Vitali

Davico, De Angelis, De Gregorio, Dell'Utri,